L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

nella seduta antimeridiana del 15 aprile è proseguita la discussione generale.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in quest'Aula per esprimere le considerazioni del Governo relativamente al disegno di legge di riforma dell'avvocatura

di regole e di funzionamento dell'avvocatura italiana. Alla fine di agosto del 2008 ho convocato al Ministero della giustizia i presidenti degli ordini del comparto giuridico-economico, nell'ambito di coloro i quali, tra gli ordini, sono sottoposti al controllo e alla vigilanza del Ministero della giustizia, e ho chiesto loro di impegnarsi a riflettere su quali potessero essere gli elementi di modernizzazione della professione forense che, senza contraddire i passi in avanti compiuti in questi anni, potessero davvero far svoltare la professione forense. Gli ordini forensi hanno approfondito tale tematica, hanno tenuto innumerevoli riunioni nel corso dei mesi e sono arrivati per la prima volta ad una soluzione testuale di ipotesi normativa, che è stata consegnata al Parlamento e che molti parlamentari e molti Gruppi parlamentari hanno appoggiato. il Governo ribadisce in questa sede la condivisione dell'impianto, la rivendicazione del metodo e l'origine prima del provvedimento che nasce da quell'incontro dell'agosto 2008, cui hanno fatto seguito - intendo ribadirlo - laboriosi ed intensi incontri tra i rappresentanti di tutti gli ordini territoriali dell'avvocatura italiana. È evidente che l'attuale disciplina forense, risalente all'ormai lontano 1933, è unanimemente avvertita come non più adeguata, per un verso, a soddisfare l'imprescindibile esigenza di attuare il fondamentale principio costituzionale del diritto di difesa del cittadino e, per altro verso, a consentire uno svolgimento delle stesse attività professionali rispondente ai requisiti di dignità e decoro che devono presiedere alle delicate funzioni dell'avvocato. La riforma dell'ordinamento forense deve segnare, a nostro avviso, il primo passo di un più ampio progetto di riordino dell'intero comparto delle libere professioni, innanzitutto degli interessi dei cittadini che verranno tutelati, puntando a garantire con più rigore la qualità del prodotto professionale; essa costituirà il punto di equilibrio tra la tutela del consumatore cittadino, la tutela della dignità dei professionisti, la garanzia di un futuro dignitoso ai giovani meritevoli ed il rispetto degli impegni comunitari. Pensiamo di poter individuare un punto di equilibrio nell'ambito della riforma delle professioni tra questi quattro obiettivi. È importante che tale ampio disegno di riforma prenda l'abbrivio dal provvedimento oggi in esame, anche per il forte valore simbolico della professione dell'avvocato, tesa a garantire alla società in cui questi opera il rispetto dei diritti fondamentali, lo Stato di diritto e la sicurezza nell'applicazione della legge. Questo intervento legislativo, come gli altri che il Governo intende varare a breve, pone rimedio ad un errore di fondo che accomuna tutti gli interventi del precedente Governo L'errore consiste nell'aver contrapposto gli interessi dei professionisti a quelli dei cittadini, immaginando questi interessi come antagonisti, immaginando cioè che l'interesse del cittadino-consumatore fosse contrapposto ed antagonista a quello del professionista, senza considerare che il professionista, erogatore di prestazioni nel proprio campo, è fruitore di servizi in tutti gli altri e quindi è a sua volta cittadino e consumatore. Questo metodo ci ha consentito di ribadire che l'unico vero e grande tesoro che l'avvocato può accumulare nell'ambito della sua carriera non è economico, ma consiste fondamentalmente nella fiducia e nella stima del suo cliente, che sceglie di andare dal suo avvocato riponendo nelle mani dello stesso i beni più preziosi come la libertà, l'onore e financo i sentimenti familiari. Dobbiamo quindi ripartire da ciò: dal fatto che il legame tra il cittadino e l'avvocato è basato essenzialmente sulla fiducia e che questo prezioso affidamento va preservato e tutelato da ogni possibile abuso. Non possiamo peraltro dimenticare quel che ci rammenta l'Europa, e cioè il fatto che il settore delle professioni è insitamente caratterizzato da un'evidente asimmetria informativa: i professionisti dispongono di un elevato livello di competenze tecniche che i consumatori non necessariamente possiedono, sicché questi ultimi incontrano difficoltà per valutare in senso tecnico la qualità dei servizi loro prestati. Ecco perché è indispensabile, per tutelare davvero il cittadino-consumatore, responsabilizzare al massimo gli ordini professionali, rendendoli i primi garanti della qualità dei servizi resi dai loro iscritti ed allontanando qualunque tentazione di corporativismo. L'avvocatura italiana - gliene do atto - ha saputo cogliere per prima il segno di questa ineluttabile evoluzione ed è stata capace di ritrovare la sua unità su questo disegno di legge, che ha visto la condivisione, come dicevo poc'anzi, di tutte le più svariate sensibilità dell'avvocatura italiana. Si inquadrano nel segno di un'inequivocabile maggiore tutela del cittadino importanti novità come l'introduzione dell'obbligo di aggiornamento professionale degli avvocati, la possibilità di riconoscere dei titoli di specializzazione attraverso appositi esami, l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile dei professionisti. Ugualmente va per intero condivisa la riforma del sistema degli albi, con l'introduzione della necessità della prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione al fine di mantenere l'iscrizione nell'albo degli avvocati e con l'eliminazione dell'iscrizione automatica all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ad oggi possibile con il solo requisito dell'anzianità. Tali importanti innovazioni garantiranno una maggiore affidabilità degli albi, impedendo iscrizioni meramente formali e consentiranno soltanto ai professionisti più valenti la difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori, eliminando un automatismo foriero di conseguenze negative in primo luogo per i cittadini, e cioè per l'utenza. Del pari fondamentale appare la riforma del sistema disciplinare, con la differenziazione dell'organo inquirente, responsabile dell'istruttoria disciplinare, da quello giudicante e con l'introduzione dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare, oggi soggetta ad una discrezionalità che alimenta, seppur talvolta ingiustificatamente, sospetti di forte corporativismo. Il Governo condivide - vi sarà già stato chiaro - la struttura portante del disegno di legge e prende atto del largo consenso formatosi sul testo oggi in discussione. Per questo motivo ha finora sostenuto l'attuazione di di questo disegno di legge e l'intenzione riformatrice, rimettendosi alla saggezza del Parlamento per operare le modifiche, secondarie, necessarie per un ulteriore affinamento del testo. Siamo consapevoli del fatto che alcuni aspetti di questa riforma meritano un approfondimento, che il dibattito parlamentare, ne siamo certi, saprà assicurare nel modo migliore. Abbiamo apprezzato la modifica introdotta nell'ambito dei lavori parlamentari in Commissione giustizia qui in Senato che ha restituito al Ministero della giustizia, in via generale, il potere regolamentare in materia di ordinamento forense. Va ricordato infatti che il potere regolamentare costituisce diretta derivazione del potere di vigilanza esercitato dal Ministero del quale ho la responsabilità su tutti gli ordini professionali ed è un potere strettamente connaturato alla natura pubblicistica del sistema ordinistico, così come sancito dall'articolo 33 della nostra Carta costituzionale. Il Governo auspica che venga rapidamente trovato un giusto punto di equilibrio tra il diritto di accesso alla professione da parte di tutti in condizioni di parità, sia formale che sostanziale, con un maggiore rigore nella selezione degli aspiranti. Appare altresì indispensabile incrementare le possibilità di scambio culturale con altre libere professioni grazie alla possibilità di creare società multidisciplinari di professionisti, e nel fare ciò il mondo dell'avvocatura, come tutti i liberi professionisti odierni, è chiamato ad un particolare sforzo di lungimiranza per evitare che modelli normativi troppo rigidi possano ostacolare una effettiva competitività a livello europeo. La necessità poi di garantire anche la trasparenza dei rapporti con i clienti impone un'importante semplificazione della disciplina delle tariffe professionali, per renderle semplici, eque e comprensibili ai cittadini. Le tariffe professionali non possono più rappresentare un labirinto: devono diventare un rettilineo. Sul punto è forte la richiesta da parte del mondo delle professioni della reintroduzione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari. Al riguardo, le iniziative assunte dal precedente Governo, sebbene adottate sotto la bandiera della tutela dei consumatori, non hanno apportato, a nostro avviso, alcun apprezzabile beneficio per i consumatori medesimi, mentre hanno danneggiato fortemente i professionisti, privandoli di una fondamentale tutela proprio nel momento in cui si abbatteva su di loro la crisi. La riforma della professione forense dovrà, al riguardo, sancire un binomio inscindibile tra la qualità elevata della prestazione e l'adeguatezza del compenso. Non possiamo più negare ai liberi professionisti il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa, che deriva da una retribuzione realmente proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto. Da questo punto di vista, svolgo una riflessione supplementare. In pura teoria tutti siamo favorevoli alla tariffa più bassa; altrettanto vero però è che alla tariffa più bassa non può corrispondere un più basso livello di aggiornamento professionale, un più basso livello di informatizzazione dello studio, un più basso livello di qualità deontologica della professione, un più basso livello di qualità e di quantità di investimenti nello studio professionale. Ecco perché il punto di equilibrio non è banale, e non si può immaginare che la sola bassa tariffa di per sé sia il sistema più efficace per garantire la qualità del servizio e il migliore servizio al cittadino, se non vi è una sistema di regole che assicuri che il cittadino venga proprio tutelato in termini di qualità del servizio professionale reso. A monte del tema della obbligatorietà delle tariffe vi è la ben più grave questione della correlazione tra qualità della prestazione professionale e quantità del compenso in via più generale, poiché non possiamo consentire che, sotto l'egida di principi in astratto condivisibili, si verifichino corse al ribasso delle parcelle, con conseguente compromissione della qualità delle difese e, conseguentemente, dell'effettività dei diritti dei cittadini. Il disegno di legge che si trova oggi sottoposto alla vostra attenzione, onorevoli senatori, ambisce a diventare una disciplina volta ad assicurare l'indipendenza, la competenza, l'integrità e la responsabilità degli avvocati italiani, garantendo al contempo la qualità dei servizi da loro resi. La competitività del nostro Paese, in termini sia di capacità di attrarre investitori, e anche capitali, sia di difendere il livello di vita dei cittadini e dei residenti in Italia, non può che passare per un sistema di giustizia più efficiente e al passo con i tempi. L'avvocatura italiana ha deciso di accettare la sfida lanciata dal nostro Governo per una giustizia più efficiente ed ha chiesto di essere dotata di strutture organizzative e di regole professionali più moderne. L'Italia ha bisogno di un'avvocatura più moderna, più aperta alle esigenze di una società multiculturale e di un'economia transnazionale e, al contempo, in grado di rispondere con efficienza e professionalità ad una domanda di giustizia sempre più ampia. Il disegno di legge di riforma dello statuto dell'avvocatura oggi in discussione appare idoneo ad assicurare il raggiungimento di tali importanti obiettivi. Per questa ragione il Governo non ha inteso presentare fino ad ora proposte emendative, ritenendo di poter procedere al superamento delle perplessità poche, invero, per quanto ci riguarda - poste dal provvedimento sia sul piano formale che sostanziale in sede di esame delle proposte emendative parlamentari. Riteniamo che sia necessaria una meditazione sul tema della riserva esclusiva in favore degli avvocati delle delle attività di assistenza, difesa e consulenza legale, soprattutto in considerazione della concorrente necessità di apprestare strumenti idonei a garantire la consulenza legale anche ai cittadini non abbienti. Appare auspicabile un punto di equilibrio ancor più ponderato in riferimento ai criteri attraverso i quali dovranno essere valutate effettività e continuità dell'attività lavorativa per il mantenimento dell'iscrizione nell'albo degli avvocati e delle modalità di riconoscimento delle specializzazioni. Attenzione particolare merita ancora il tema del tirocinio professionale in considerazione del fatto che per consentire il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi che questa riforma si prefigge andranno efficacemente contemperati il rigore nella selezione dei professionisti con il diritto di tutti ad accedere all'albo in condizioni di parità. Siamo tuttavia convinti che la saggezza del Parlamento saprà trovare il giusto contemperamento tra contrapposti interessi in gioco ed auspico fortemente che questa riforma giunga in tempi rapidi all'approvazione del Parlamento. L'innalzamento del livello della professionalità dell'avvocatura è uno strumento indispensabile per garantire l'efficienza del sistema giudiziario del nostro Paese e per combattere il cancro dell'eccessiva durata dei processi; e senza la collaborazione fattiva del ceto ceto forense qualsiasi volontà riformatrice, per quanto determinata, rischierebbe il fallimento. Ecco perché noi ci stiamo sforzando di condurre in porto un disegno di legge che restituisca all'avvocatura la sua originaria missione, che è quella di una vocazione. Noi con questo disegno di legge stiamo compiendo un grande sforzo che passa dalle modalità di accesso al modo per rimanere avvocati, al modo per difendere in Cassazione, che l'avvocatura non debba e non possa più essere la strada del laureato in giurisprudenza che non ha altre strade *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Mazzatorta)*, la strada del laureato in giurisprudenza che non ha altri sbocchi, lo sbocco del laureato in giurisprudenza che non vince altri concorsi. L'avvocatura è una vocazione; l'avvocatura deve essere posta al servizio dei cittadini, e speriamo con questo disegno di legge di fare un importante passo avanti in questa direzione.

Signora Presidente, approfitto della presenza del Ministro in Aula ancora per qualche minuto per ricordargli che la deputata radicale Rita Bernardini è giunta, assieme a dirigenti e militanti radicali, al settimo giorno di sciopero della fame per richiedere quello che è stato annunciato più volte dal Governo, cioè un provvedimento relativo alle scarcerazioni: qualcosa di assolutamente urgente che, se come già accaduto in passato - si riesce a trovare la consonanza di maggioranza e alcune parti dell'opposizione, si può tecnicamente guadagnare con poco tempo. Ripeto: un membro del Parlamento è in sciopero della fame insieme a decine di persone da sette giorni per chiedere

Spero quindi che, anche a seguito di questo appello, il Ministro voglia prendere in considerazione ogni possibilità per accelerare questo processo decisionale. In passato, i radicali hanno sempre avuto grande vicinanza all'avvocatura italiana, in particolare negli anni '80 per le battaglie denominate di "giustizia giusta": una giustizia che voleva porre al centro i diritti individuali, e che ha elaborato, proprio grazie alla partecipazione attiva di molti avvocati italiani, e in particolare dei rappresentanti delle camere penali, tutta una serie di proposte, che si sono tradotte a volte in *referendum*, a volte in iniziative parlamentari e, buone ultime, in una serie di mozioni fatte proprie da questo Governo nel 2008, nel 2009 e nel 2010 relativamente alla riforma della giustizia: una riforma della giustizia che vuole abolire l'obbligatorietà dell'azione penale, che vuole separare le carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante e che vuole reintrodurre quanto i cittadini italiani 25 anni fa avevano deciso attraverso un *referendum*, cioè la responsabilità civile del magistrato. Questa collaborazione, direi pressoché quotidiana, con gli avvocati italiani ci ha portato anche, ogniqualvolta i radicali hanno tenuto un loro congresso, ad avere all'interno del congresso, una commissione sulla giustizia, o meglio sulla malagiustizia

e le sentenze pressochè quotidiane che la Corte europea dei diritti umani emette contro il sistema Italia di amministrazione della giustizia. Ma proprio quella vicinanza, quella lotta comune con gli avvocati ci ha portato all'ultimo Congresso, quello che si è tenuto a Chianciano dal 12 al 15 novembre 2009, ad adottare una mozione particolare - prima firmataria, per l'appunto, un giovane avvocato, Deborah Cianfanelli, membro di Radicali italiani - che è stata fatta propria dal Congresso e che mi appresto a leggere: il disegno di legge n. 1198 per la riforma forense non costituisce una riforma della professione, volta a recepire le esigenze e le difficoltà segnalate da chi la professione esercita, ma è un vero e proprio tentativo di ritorno spudorato alle corporazioni, col chiaro obiettivo di serrare i ranghi dell'ordine attraverso la previsione di una serie molto incisiva di limiti e requisiti sia per l'accesso che per l'esercizio della professione di avvocato».

Le principali restrizioni sono: 1. Forti restrizioni sia all'accesso che all'esercizio della professione: viene infatti previsto un *test* obbligatorio per poter iniziare il tirocinio della durata di due anni, con contestuale obbligo della frequenza di corsi di formazione organizzati, ovviamente, dai consigli dell'ordine. In questo modo viene a svilirsi la formazione conseguita con gli studi universitari; viene inserito inoltre il limite dell'età di 50 anni per l'ammissione all'esame di abilitazione. 2. Rigidi requisiti per la permanenza nell'ordine professionale: la permanenza dell'iscrizione all'albo viene subordinata all'esercizio effettivo e continuativo della professione, la cui sussistenza è desumibile presuntivamente anche dalla percezione di un livello minimo di reddito. Sotto la soglia minima di reddito non si è avvocati e l'Ordine disporrà la cancellazione dall'albo, trasformandosi così anche in controllore fiscale. Questo a scapito delle categorie più deboli ossia dei giovani professionisti che faticano ad affermarsi con un proprio "parco clienti", sia, ad esempio, delle donne che sono costrette a sospendere l'attività lavorativa per gravidanza e non riescano a conseguire per un paio d'anni la soglia minima di reddito o a coprire i requisiti di continuità richiesti. 3. Modifica della disciplina dell'accesso alle giurisdizioni superiori: diminuiscono da 12 a 10 gli anni di esercizio della professione richiesti agli avvocati per patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma gli anni di carriera alle spalle non basteranno più, da soli, a legittimare l'avvocato dinanzi alle corti superiori, ma sarà necessaria la frequenza, con profitto, di una Scuola superiore dell'Avvocatura che il CNF è delegato ad istituire e regolamentare». Questo, per quanto riguarda il merito, riteniamo che dia adito a qualcosa di più di quanto detto poc'anzi dal Ministro, e cioè a delle «perplessità»: crea enormi problemi dal punto di vista di quello che, mi pare molto ingenerosamente, il Ministro poc'anzi ha chiamato essere stata la decisione dello scorso Governo Prodi, quando, grazie ad una serie di liberalizzazioni promosse dall'allora ministro Bersani, secondo l'interpretazione del ministro Alfano si sarebbe andati a mettere in contrapposizione gli interessi dell'utente con quelli del professionista. Ebbene, no: qui si fa il ragionamento inverso, ed il merito, denunciato da tutti gli interventi in discussione generale e, sono certo, anche da quelli che seguiranno questo, si unisce in maniera molto preoccupante al metodo con cui si è arrivati a preparare questo disegno di legge. L'ha ricordato poc'anzi anche il Ministro: tutto, o buona parte, scaturisce da una riunione tenutasi nell'agosto 2008 tra i rappresentanti di categoria. In qualche modo si è dato pieno titolo non di suggerimento, ma di vera e propria preparazione di una legge, all'Ordine che deve rappresentare i professionisti che ne fanno parte. Si è più volte sottolineata la pericolosità di questo metodo di proseguire. Stiamo, infatti, parlando di una professione - la più liberale delle professioni - che deve tutelare i diritti individuali di fronte allo Stato, di fronte a tutti i possibili soprusi che le leggi dallo Stato possono esercitare nei confronti dei propri cittadini per una serie di accuse,

come a volte gli avvocati hanno fatto in passato, il problema di individuare nell'ordine stesso uno degli aspetti da scardinare per rendere la più liberale delle professioni quanto più liberale possibile, sia per quanto riguarda l'accesso sia per quanto riguarda la permanenza e l'esercizio dell'attività. L'Ordine, quindi, non diventa un garante, ma il vero e proprio comandante, non soltanto al proprio interno, ma anche nei rapporti che intrattiene con le istituzioni, istituzioni che invece dovrebbe contrastare.

Forse in Italia non esistono sufficienti processi che necessitano di assistenza legale? Forse in Italia non esistono problemi legali legati a nuove possibilità? Penso, in particolare, a tutti i diritti digitali che recentemente si stanno affermando: hanno forse bisogno di un'ulteriore offerta di assistenza legale? Tutto questo, se dovesse mai essere un problema (e io non credo che l'eccessivo numero degli avvocati in Italia sia un problema), non si affronta certamente innalzando una palizzata dinanzi a tutti quelli che vogliono accedere accedere a quella professione, ma paradossalmente aprendo quanto più possibile il mercato e consegnandolo alla dinamica della domanda e dell'offerta. È stato più volte ricordato come in altri Paesi sia consentito fare addirittura la pubblicità per far conoscere ai propri clienti che si ha un vero e proprio studio professionale. Se prendete un autobus o una metropolitana nel Nord Europa o negli Stati Uniti, vedrete che una pubblicità su due è di uno studio legale che parla, per l'appunto, di un problema che questo Governo ha voluto porre al centro del proprio pacchetto sulla sicurezza: quello dell'immigrazione. Ebbene, immaginate quante persone hanno oggi bisogno di assistenza legale, non possono permettersela e dovrebbero andare un domani a scontrarsi con una categoria che ha addirittura reintrodotto i minimi garantiti o, comunque, una soglia minima per quanto riguarda le parcelle. non riprende quello che in teoria avrebbe scompensato il Governo Prodi, e cioè l'equilibrio cioè tra i diritti degli utenti e i diritti dei professionisti, ma sbilancia dalla parte degli avvocati tutta una serie di privilegi certificati da questo disegno di legge. Spero quindi che le perplessità manifestate dal Ministro aumentino, anche a seguito del prosieguo del nostro dibattito, e spero che si voglia avviare una serie di dibattiti pubblici nei quali quali dovremo confrontarci non soltanto con la maggioranza e tutti coloro i quali all'interno del Parlamento sostengono questa proposta di riforma, ma anche con la categoria in questione, perché all'interno della stessa - e penso in particolare all'Unione dei giovani avvocati italiani - esiste un gruppo che nutre forti dubbi che questa sia una riforma piuttosto che una controriforma.

il voto che il Senato esprimerà al termine della discussione ora in corso è un voto di grande rilevanza. Si tratta di un modo di dire, naturalmente perché, in realtà grande rilevanza hanno tutti i voti che sono espressi in quest'Aula e in quella in cui siede la Camera dei deputati. Solo un modo dire, dunque, soltanto per enfatizzare il momento in cui si concluderà la prima fase del processo di modernizzazione di un sistema che è nato ben 77 anni fa che è preposto al governo delle sorti professionali di oltre 230.000 avvocati, con un indotto generato di misura attendibilmente individuabile intorno al milione, alle 750.000 persone. 230.000 avvocati alle cui cure sono affidati gli oltre 5 milioni e mezzo di procedimenti civili che risultavano pendenti alla fine del 2008, in vari gradi di giudizio, davanti ai tribunali italiani. Per non dire dei 3 milioni e mezzo (questo ci dicono i sistemi informativi del Ministero) di processi penali su cui dovranno pronunciarsi le nostre corti, per riferire solo di quelli che riguardano gli imputati noti, perché - a considerare quelli con imputati non noti - il banco salterebbe in un istante. La relazione che introduce il testo che la Commissione giustizia del Senato ha offerto all'Aula (e quanto ad essa ha aggiunto il relatore, senatore Valentino) riferisce del contributo dato alla predisposizione del testo di partenza dagli stessi avvocati, attraverso le proprie associazioni e, soprattutto, attraverso l'opera di sintesi svolta da coloro che fra essi siedono nel Consiglio nazionale forense. Si tratta di un contributo non secondario, di cui penso abbia fatto senz'altro gran bene a tenere conto la Commissione, pur senza per questo sottrarsi al dovere ed alla responsabilità della produzione di un ulteriore testo, ancora più evoluto, che è quello che è ora esaminato. Così come, del resto, dovrà ora darsi cura di fare quest'Aula, con riferimento allo stesso, e così come dovrà eventualmente essere da parte dei colleghi deputati perché alla fine risultino davvero raccolti e vagliati proprio tutti i punti di vista, di tutte le parti interessate, di tutti gli interpreti delle varie funzioni che interessano il sistema - cittadini ed utenti, anche attraverso le loro associazioni di tutela, professionisti, giudici e dottrina - nell'ottica di stabilire uno strumento che sia funzionale (ed il più possibile performante) ai prossimi anni della professione dell'avvocato. Prossimi anni che non saranno anni qualsiasi per plurime ragioni: perché nel corso degli stessi si consolideranno gli effetti e le procedure innovativamente introdotti nell'ordinamento giudiziario dalla «riforma Castelli» per quanto riguarda i suoi aspetti differiti perché nel corso degli stessi muoveranno i loro passi i frutti legislativi di quel complesso di interventi di innovazione che va sotto il nome di riforma della giustizia. Riforma della giustizia che è nell'agenda dell'attuale maggioranza e del Ministro Guardasigilli; che è secondo alcuni urgente, secondo altri indifferibile (per altri ancore forse meno); che, personalmente, mi limito a conclamare come indispensabile e inevitabile alla luce dei tempi e degli equilibri sociali mutati, alla luce del progressivo non corretto uso che della stessa è stato da molti dissennatamente fatto, e quindi nella necessità - questa sì non differibile di ripristinare quell'equilibrio istituzionale che coloro che consegnarono al Paese la vigente Costituzione ebbero a prudentemente stabilire e a sapientemente modulare, che non altrettanta successiva prudenza legislativa ha invece contribuito a sbilanciare, con la concorrente colpevole miopia di molti detentori del potere dell'informazione...

...coniugata alla inescusabile scorrettezza di molti (sempre più) che, arbitri della giustizia, si sono mostrati del tutto dimentichi del fatto che proprio il loro alto ruolo, troppo spesso non adeguatamente onorato, li ha consegnati e li consegna ad essere soggetti alla legge, soltanto alla legge: massima responsabilità, dunque, non ottusamente scambiabile per un ingiustificato privilegio. L'avvocato di tutto questo, in questi prossimi anni, dovrà essere un protagonista credibile e indiscusso, per contribuire a garantire la ritrovata efficacia del processo civile nei suoi tempi e nella sua affidabilità, fermo - come sono e come credo che tutti debbano essere - nella convinzione che si tratti dell'unico ammissibile strumento destinato a regolare i conflitti interni alla comunità (vera sconfitta, attraverso la sua funzionalità, per le società criminali dell'altro Stato), strumento creditore, come tale, anche nei confronti del legislatore, di ogni attenzione e protezione, anche in relazione alle disfunzioni sue proprie. E l'avvocato dovrà sempre più essere non solo protagonista, ma - ancor di più - pilastro centrale di un processo penale che alla garanzia di sereno e sicuro vivere per i cittadini sappia assicurare e coniugare certezza di regole, tutela di diritti e di procedure e conclusione proporzionata ed equilibrata per quanti sono ad esso sottoposti, in una stagione sociale in cui risultano non mai sopite derive giustizialiste, cui anche l'agone politico non si sottrae, e che anzi in alcuni contesti palesemente teorizza o coltiva; in un momento in cui si sentono magistrati, anche autorevoli, e giornalisti spesso intelligenti, disinvoltamente e disinibitamente impiegare nel loro dire inaccettabili definizioni, orribili nel loro inammissibile cinismo, quali quelle degli "effetti collaterali" per tentare di conferire improbabili giustificazioni ad inescusabili pervasività che sono affermate "di sistema" e che il nostro sistema mai ha, in verità, conosciuto, per essere viceversa solo banali scorciatoie da loro stessi a se stessi date, in una collisione non oltre accettabile verso valori fondanti dell'individuo (libertà, onore e onorabilità, identità e riservatezza e - perché no? - credito negli affetti familiari); in giorni in cui le cronache nuovamente riferiscono di uomini piegati da detenzioni provvisorie e protratte (ben oltre i limiti e i perimetri che la legge consente), di persone private di ogni personale futura prospettiva, non già in quanto dichiarati responsabili di crimini a seguito di processi, ma solo in quanto destinatari di anticipate risoluzioni assunte (sempre più spesso con la sapiente manipolazione mediatica del fatto) da chi è chiamato a raccogliere le prove e semmai impedire la reiterazione della condotta, e non già, certo, a rendere giustizia, in una singolare autoreferenziale solitudine (e giustizia esige, se del caso, l'irrogazione di una sanzione che appaia equa, proporzionata e pertinente, perché mai giustizia aspira invece ad uomini piegati, sviliti o privati di prospettiva di vita). L'avvocato di tutto questo dovrà continuare ad essere centrale pilastro di riferimento e di sostegno del diritto, e perché questo sia dovrà presentarsi esso stesso sostenuto e sempre più credibile, anche attraverso regole rinnovate e rese più incisive in relazione ai nuovi tempi e a più evolute opportunità. Questo è il senso della riforma che il Parlamento voterà: per una professione più efficiente, più matura, più consapevole e meno autoreferenziale. Questa è la speciale importanza che annetto al voto della nostra Ho avanzato numerose proposte emendative che i colleghi senatori vorranno valutare: alcune tendono a rimuovere qualche aporia che mi è sembrata essere rimasta nel testo; altre hanno la presunzione di meglio scrivere talune disposizioni che pure sono di centrale rilievo.

in tutte le sue articolazioni (prima fra tutte, il Consiglio nazionale forense) può dare, unitamente a quelli che dovessero derivare dal prudenziale, doppio controllo delle Commissioni parlamentari. Molte proposte emendative, dunque, che non sono tuttavia mai sintomo di distanza rispetto ad un testo che, nell'insieme e nel proposito, condivido pienamente e convintamente, e che nemmeno possono suonare a testimonianza di disagio, anche laddove affrontano temi di particolare rilievo e delicatezza, primi fra tutti quelli che riguardano l'accesso all'avvocatura e la posizione delle nuove generazioni di avvocati. La legge del 1933 ebbe una "modernità": quella di assegnare agli avvocati larghi spazi di gestione domestica dell'organizzazione della professione, al di fuori di ogni statalismo. La riforma che è ora affrontata muove in identico ed ancora più accentuato segno, come ben testimoniano i larghi poteri di autodeterminazione assegnati ai consigli dell'ordine circondariali ed al Consiglio nazionale forense, come ancor più mostra il nuovo procedimento disciplinare che, al mantenimento del suo carattere domestico, ha il pregio di coniugare garanzie, tipizzazione delle condotte, terzietà e doveroso distacco di chi è chiamato a giudicare. Gli emendamenti presentati muovono dal presupposto del dovere non derogabile degli avvocati che deve consistere in una risposta misurata e commisurata a tutto questo, scevra da autoreferenzialità e derive protezionistiche, in primo luogo, in quelle pieghe della legge che loro riserva la responsabilità e l'onere di determinare, selezionare e in definitiva scegliere i propri futuri concorrenti, oltre che di consentire la crescita - in regime di libera e corretta competizione professionale - dei più giovani fra di loro, nell'interesse da ultimo dei cittadini, del cliente, intorno alla cui protezione il sistema - che è e deve restare "civicocentrico" - deve continuare a ruotare. in un'epoca economica in cui si allargano le lame della forbice: da una parte - vivaddio! - un rilevante maggiore tasso di scolarità che produce nuovi laureati, dall'altra un sistema pubblico che, anche complici le sopravvenute tecnologie, non assorbe più i volumi di occupati di un tempo e a cui si accompagna un'impresa privata che sempre più sfoltisce i ranghi dei propri addetti e che, spesso priva della capacità di creare nuovo prodotto, trova rapido, economico e conveniente cercare di impadronirsi di quello che c'è già e che è costituito dai saperi dei professionisti. In una tale epoca nessuno può revocare in dubbio l'enorme contributo sociale dato dalle libere professioni nell'assorbire quanti si sono presentati alla necessità di lavoro, ma è ora evidente la necessità di nuove regole che scrivano anche non tanto la protezione dei liberi professionisti (degli avvocati fra questi, in questo caso), quanto quella di un sistema che tutti gli osservatori indicano ormai unanimemente come vicino al rischio di implosione. Un tale rischio finirebbe invero per colpire non già una semplice categoria, ma piuttosto un non rinunciabile catalogo di diritti e di protezioni di tutti i cittadini. Di qui, dunque, un accesso alla professione di avvocato che rechi oggettiva selezione, ma che non sia acritico sbarramento, così come mi sono sforzato di proporre negli emendamenti in tema, e che possa parallelamente condurre a maggiori qualità e più vivaci competitività. ho ascoltato gli interventi chi colleghi che hanno diffusamente trattato tali temi in relazione all'ormai *vexata* *quaestio* delle tariffe minime e che lo hanno fatto evocando la suggestione della restaurazione. Premetto che considero benvenuta per principio qualsiasi restaurazione volta a riparare i guasti recati da incomprensibile sudditanza, soprattutto per un partito che ha la storia politica di quello che se ne è reso protagonista, protagonista, nei confronti di poteri forti, anzi fortissimi, peraltro reduci dall'inimmaginabile capolavoro dell'aver messo in ginocchio finanziariamente ed economicamente larga parte dal pianeta. Premesso ciò, mi riservo di nuovamente intervenire sul punto per svolgere qualche riflessione e soprattutto per consegnare all'Aula documentate informazioni sul punto, ma lo farò in sede di illustrazione degli emendamenti che lo trattano. Ho concluso, signora Presidente. Mi permetta solo di anticipare ai colleghi, già da ora, le mie scuse per il gran numero di emendamenti che ho proposto, anche se sono convinto che ne potrà essere assai rapida la trattazione. Mi scuseranno più facilmente se solo penseranno che è in discussione una legge di riforma della professione che ha assicurato alla mia famiglia e a me, per più decenni, un dignitoso livello di vita e alla quale credo sia forse

per conoscere la sua opinione, importante per permettere al dibattito di essere il più proficuo possibile, così da arrivare ad un testo largamente condiviso. Vede, noi dell'UDC condividiamo appieno l'esigenza di riordino del mondo delle professioni di cui il Ministro si è fatto interprete: da tempo ne abbiamo denunciato l'urgenza. La cornice normativa che disciplina alcune professioni e lascia scoperte altre non è più adeguata all'attualità e ne penalizza, tra le altre cose, lo sviluppo in senso liberale, in un quadro attualmente anche le libere professioni subiscono i contraccolpi della crisi senza avere ottenuto fino ad oggi adeguata attenzione da parte del Governo. Tuttavia, se quella forense deve rappresentare l'avanguardia di questo processo di riforma che dovrà coinvolgere tutto il mondo delle libere professioni, ebbene, dobbiamo puntualizzare alcune cose sul metodo e sul merito con cui si vuole addivenire a questa riforma pilota e, se questa ne è un'esemplificazione, su tutto il processo riformatore, convinti che in questa fase storica il nostro Paese necessiti più che mai di strumenti per aumentare la competitività al fine di promuovere lo sviluppo, per conformare la legislazione alla realtà sociale ed economica del presente uniformandola a quella di di altri Paesi europei. In quest'ottica, se una critica c'è da fare a tale riforma è che essa ha oscillato tra accelerazioni e colpi di arresto dettati dall'esigenza del Governo di dare qualche segnale in merito alla riforma della giustizia e, contestualmente, di accreditarsi come interlocutore di un'ampia categoria di professionisti senza che fino a questo momento l'Esecutivo formulasse una proposta in merito alla stessa. Ebbene, ciò che ci sta a cuore è l'autonomia e l'indipendenza del Parlamento nello scrivere le leggi, al fine di perseguire l'interesse generale, nel caso di specie a tutela della promozione e dell'affidamento della collettività sulla qualità e correttezza delle prestazioni forensi. In tal senso, si evidenzia nel testo ancora una potestà regolamentare in capo al Consiglio nazionale forense per importanti aspetti della professione. Questo organo deve essere ascoltato quale interlocutore essenziale, insieme agli altri organismi rappresentativi dell'avvocatura, per il confronto a livello istituzionale nella produzione normativa dei regolamenti che sono funzionali ad una migliore organizzazione dell'attività forense, ma lasciare che larga parte delle disposizioni regolamentari sia scritta al di fuori del Parlamento, riducendo l'organo legislativo a mera istanza di ratifica, mi sembra, proprio in ossequio a quel principio che invochiamo ed applichiamo nel rapporto con la magistratura, eccessivo e sbilanciato. Da questo punto di vista, è chiaro che il testo ci appare squilibrato. Per quanto riguarda il merito, siamo convinti che occorra adoperarsi nel non facile tentativo di conciliare modernità, concorrenza globalizzata, liberalizzazione della professione con la dignità e il prestigio della stessa. Quella dell'avvocato è, prima di tutto e al di sopra di tutto, una funzione costituzionale: egli garantisce il diritto alla difesa. Non partire da questo presupposto vuol dire non solo mortificare la professione, ma anche non dare attuazione ad un impianto costituzionale che regola l'esercizio l'esercizio della giurisdizione, e quindi sottrarre al cittadino la garanzia di principi fondamentali. Questa alta funzione va assicurata e salvaguardata anche di fronte alla pur necessaria riforma in senso liberale della professione che non può non tenerne conto e custodirne l'esercizio nelle mani di soggetti preventivamente selezionati per la loro capacità professionale e sottoposti ad un rigoroso vincolo deontologico (di trasparenza e di correttezza) e ad un controllo permanente. va confermata in seno ad un agognato riordino organico del comparto giustizia che dovrebbe camminare di pari passo. da bilanciare la parte della trasparenza cui si va incontro. Partendo da tale assioma, dopo oltre 75 anni, non possiamo non riconoscere l'urgenza di una riforma che aggiorni la cornice regolamentare della professione a nuove sopravvenute esigenze, come del resto già fatto dalle maggiori legislazioni europee, e concorra a superare una fase patologica in cui essa versa anche a causa di questo ritardo. Sono infatti tanti gli iscritti agli albi professionali degli avvocati e tale numero tende vistosamente a crescere ogni anno. Tuttavia all'aumento dell'offerta e della concorrenzialità in termini economici non corrispondono sempre una qualità e una correttezza della prestazione, conformi ad una funzione costituzionalmente rilevante che l'attività forense dovrebbe garantire. Alla riconosciuta molteplicità di problematiche (certo, di non facile soluzione) che attraversa il mondo forense questo testo non risponde, a nostro avviso, nella maniera più adeguata. Esso sembra caratterizzarsi per una serie di chiusure, denunciate, non ultimo, anche dall'*Antitrust*; mi riferisco, tra le altre, agli ostacoli frapposti all'accesso alla professione. Non possiamo non condividere le forti perplessità che i giovani avvocati e chi intende affacciarsi all'esercizio di questa attività professionale nutrono nei confronti della proposta, riguardo rispettivamente alla permanenza di iscrizione all'albo subordinatamente all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo continuativo e all'accesso. Viene introdotta una serie di barriere e limiti nello svolgimento della pratica. Mi riferisco, in particolare, al test di ingresso che si istituisce per la mera iscrizione all'albo. Inoltre, si rende incompatibile l'esercizio del tirocinio con qualsiasi rapporto di impiego pubblico, con l'esercizio dell'attività di impresa e con lo svolgimento di altri tirocini. Se a ciò si somma che nel provvedimento non si prevede alcun tipo di remunerazione o compenso per il praticante, anzi si precisa precisa che lo svolgimento del tirocinio non comporta comunque l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato, in senso peggiorativo rispetto a quanto previsto attualmente nel codice deontologico, si comprende come si vogliano istituire

Ciò risulta eccessivamente rigido rispetto alla necessaria flessibilità che dovrebbe caratterizzare un periodo prodromico ed incerto rispetto all'effettivo esercizio della professione che potrà essere espletata solo con il conseguimento del titolo. Al contrario, avremmo salutato con favore la proposta di svolgere la pratica già durante il corso universitario o la previsione di forme di sostegno, quali borse di studio a favore dei tirocinanti, in modo da garantire a tutti l'accesso. Siamo convinti che i tempi e soprattutto i costi dell'espletamento di un periodo che di fatto posticipa l'ingresso nel mondo del lavoro debbano essere ridotti. Ulteriore aspetto di perplessità riguarda l'attività stragiudiziale. Esiste un solo motivo per cui la consulenza stragiudiziale, l'assistenza giuridica che non comporta accesso alle aule giudiziarie, debba essere riservata soltanto a chi è iscritto all'albo degli avvocati? C'è un solo motivo per cui non possa esprimere un proprio parere su una qualsiasi questione giuridica un esperto in quel settore non perché avvocato, ma perché se ne è occupato comunque in modo continuativo e professionale? Inoltre, la proposta in esame riformula il novero delle incompatibilità degli avvocati ampliandone la portata, vieta espressamente la costituzione di società di capitali e prevede che l'associato o il socio possano far parte di una sola associazione. Il funzionamento del sistema delle specializzazioni, poi, è lasciato alla disponibilità esclusiva del Consiglio nazionale forense. Questo non può non destare dubbi di natura concorrenziale. In tema di pubblicità, nell'era del mercato globale questa proposta limita la comunicazione sull'offerta legale alla targa appesa alla porta dello studio. L'opportuna norma che prevede l'obbligo dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione entrerà in vigore contestualmente e secondo i contenuti di non meglio precisate direttive comunitarie in corso di emanazione, e quindi, di fatto, è svuotata del suo contenuto. Un altro aspetto su cui voglio porre l'attenzione è poi quello particolarmente sensibile che riguarda le tariffe. A distanza dalla loro introduzione, non possiamo non riconoscere come le cosiddette lenzuolate dell'onorevole Bersani non abbiano prodotto alcuni degli effetti auspicati; tuttavia non ci convince il mero ritorno all'inderogabilità dei minimi tariffari e alla contestuale derogabilità dei massimi prevista dalla proposta. Quello di cui siamo certi è che le tariffe, così come sono, risultano inadeguate soprattutto a soddisfare l'esigenza di trasparenza e di chiarezza giustamente invocata dai cittadini. Ridurre la questione alla reintroduzione o meno dell'inderogabilità dei minimi tariffari mi pare una disputa ideologica e riduttiva del problema. Siamo lungi dal dire che siamo di fronte ad una riforma facile, su cui sarà semplice giungere ad un indiscusso consenso. Su di essa si concentrano molte aspettative e ritardi maturati nel corso di oltre 75 anni di attesa. Essa deve contemperare molte esigenze non facilmente conciliabili: deve consentire di attuare pienamente il diritto alla difesa, ma deve anche preparare questa libera professione, così rilevante, ad applicare le regole della concorrenza indicate dalle norme comunitarie, pur nel rispetto della deontologia e dell'offerta di un qualificato servizio ai cittadini. Lo deve fare, a nostro avviso, rispettando queste linee guida: coordinare la nuova disciplina con quella comunitaria; evitare che crescano ulteriormente i costi a carico dei cittadini nel ricorso alla giustizia, come invece ha denunciato l'*Antitrust*; prevedere una normativa innovativa per l'accesso alla professione che garantisca un'appropriata selezione dei molti aspiranti ed un'adeguata formazione dei nuovi avvocati e che tuttavia non mortifichi le capacità e le aspirazioni dei più giovani; imporre poi un'elevata professionalità a tutti gli iscritti con un obbligo costante di aggiornamento di tutti, anche di coloro già all'interno degli ordini, senza esclusione alcuna.

dopo tanti anni di agognata attesa, l'interesse è che si arrivi ad una riforma che soddisfi le aspettative e duri nel tempo, nell'interesse generale del Paese.

è stato detto da più parti che questa riforma è attesa, ed è vero, da oltre settant'anni. Uno spazio temporale lunghissimo entro il quale abbiamo registrato profonde trasformazioni economico-sociali, cambiamenti epocali indotti dai moderni strumenti di informazione e comunicazione, l'introduzione nel nostro ordinamento di princìpi e norme comunitarie sulle professioni libere, sulla liberalizzazione dei mercati dei servizi e dunque il ruolo dell'avvocato nella società italiana è profondamente mutato. Eppure, la legge sull'ordinamento forense era ed è rimasta la stessa. Vi è quindi la necessità di approvare questa riforma e su questo concordiamo, e non da oggi. Una riforma importante. Il lavoro della Commissione, come ha detto il relatore, senatore Valentino, è stato approfondito, approfondito, apprezzabile, uno sforzo importante di sintesi che si è rivelato più difficile di quanto potesse apparire

diversi, alcuni dei quali vengono in maggiore evidenza nella fase cruciale, quella della discussione in Aula. Comunque, da qualche parte bisognava collocare il punto di equilibrio tra le varie scelte possibili

possibile, seppure dentro una cornice di difficoltà nell'operare delle scelte. Siamo sicuri che non è possibile fare qualche passo ulteriore verso una migliore sistemazione dei punti cruciali del provvedimento?

possa dare qualche risposta positiva nel corso dell'esame del provvedimento. Certo, per alcuni aspetti l'equilibrio trovato è assolutamente condivisibile, per altri, a mio modo di vedere, non lo è e c'è bisogno di un ulteriore intervento in Aula. Ci sono ampi margini di miglioramento e d'altra parte l'esame dell'Assemblea deve servire proprio a vagliare l'esito del confronto che si è tenuto nella Commissione di merito, apportando le modifiche ulteriori che riterremo necessarie nell'ambito di un confronto che mi auguro continui ad essere costruttivo. Ho apprezzato molto, ad esempio, lo spirito, oltre che una parte del contenuto,

il tema del praticantato e dell'accesso. Si è discusso molto di questo argomento in Commissione e se ne discute anche nel Paese

Purtuttavia, noi non possiamo accettare, credo, che per poter soddisfare questa esigenza, quella di maggiore rigore e maggiore selettività nella fase di praticantato e di accesso alla professione, si penalizzi - a me sembra - in modo molto serio la possibilità per i giovani meritevoli di accedere fruttuosamente all'esercizio di questa importante professione. Mi riferisco all'incomprensibile

delle specializzazioni: mentre gli avvocati che già esercitano da dieci o venti anni hanno un canale di accesso alle specializzazioni, i giovani, invece, i giovani, invece, devono sottoporsi ad un *iter* complesso per poter conseguire il titolo specialistico, oltre che per poter accedere alle magistrature superiori.

anche alla necessità di una presa d'atto normativa e di una migliore sistemazione legislativa della realtà attuale degli uffici legali in Italia, laddove gli avvocati giovani, i praticanti, ma anche gli avvocati titolati, svolgono funzioni a funzioni a volte assimilabili a quelle di un lavoratore dipendente. È dunque giustificata la contrarietà dei giovani (non solo dei giovani avvocati) alla sistemazione normativa proposta dalla Commissione? Penso di sì, e penso anche che si possano dare risposte diverse, non mettendo in discussione

accedano coloro che hanno professionalità, titolo, preparazione per poter esercitare una professione così importante. Penso, pertanto, che si debba assolutamente eliminare la previsione della prova preselettiva, che si debba rivedere il regime delle incompatibilità nella fase del praticantato, che si possa intervenire sulle tariffe minime a vantaggio dei giovani avvocati

Vi chiedo perdono se faccio un esempio personale. Io sono diventato avvocato, e mi onoro di appartenere all'avvocatura e di avere esercitato questa professione

il figlio di una famiglia di genitori poco agiati si possa permettere per 8-10 anni di non percepire alcun reddito per poter accedere, appunto, all'avvocatura? Non è possibile e non possiamo non possiamo penalizzare in modo - consentitemi l'utilizzo di un termine antico - classista i giovani del nostro Paese. Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo modificare queste norme. Vi è poi il tema delle società, che ha a che fare con la modernità dell'esercizio di questa professione e con il modo con il quale gli avvocati stanno nel mercato dei servizi professionali non solo del nostro Paese, ma anche dell'ambito europeo

forense, nonché società o associazioni professionali multidisciplinari, in cui - non è detto, ma si presume che sia così - l'attività forense sia prevalente rispetto all'esercizio di altre attività, ed introduce l'ipotesi

avvocato. Trovo alquanto discutibile e contraddittorio che, da un lato, si ampli in modo, a mio parere, eccessivo la riserva di esclusiva dell'esercizio della professione forense per ogni tipo di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e, dall'altro, si consenta che nel nostro Paese si possa esercitare la professione di di avvocato anche da parte di società magari composte da cinque architetti, tre ingegneri, due commercialisti e un avvocato, in tal modo svilendo la dignità e le caratteristiche proprie dell'esercizio della professione forense. Così come ritengo che si sia trattato in modo eccessivamente liquidatorio il tema delle società di capitali. Conosco gli argomenti che vengono addotti, gran parte dei quali condivisibili, contro l'ipotesi che, contrariamente a quanto avviene in molti altri Paesi europei, si possa esercitare la professione forense a mezzo di società di capitali, ma credo che si possa compiere uno sforzo:

perché non era possibile introdurre norme di quel tipo in modo avulso da una riforma più organica delle professioni e, nel nostro caso, della professione forense. È vero che grandi *lobby*, come diceva il collega Caruso prima, hanno utilizzato per loro convenienza

ben note cause seriali, che prevedono che l'avvocato faccia la fotocopia di una causa identica per centinaia o migliaia di volte chiedendo per ciascuna di esse il minimo tariffario?

confrontarsi per dare una risposta alle molte osservazioni, talune anche assai polemiche, anche se più nelle sedute precedenti se più nelle sedute precedenti che non stamattina, che abbiamo avuto modo di ascoltare. Intanto, mi permetterete di dire, in relazione a quello che sentii nella prima seduta dedicata alla discussione generale,

perché in relazione a questo proprio non ve ne sono. Sarò l'ultimo in questa Aula ad andare a speculare sulle differenti sensibilità o su pensieri non esattamente l'uno all'altro sovrapponibili. Questo Questo è un Parlamento, e ci mancherebbe altro che andassimo a speculare sulle differenze di mentalità e sulle diverse sensibilità nell'approccio ad argomenti privilegiati che possono essere in capo all'uno o all'altro.

che ben altra è la posizione dell'Italia dei Valori come manifestata, ad esempio, dall'illustre senatore Li Gotti che - non voglio minimamente interpretarlo, non me ne prendo la libertà - è sostanzialmente d'accordo su alcuni capisaldi informatori della riforma e, comunque, è d'accordo su punti qualificanti della medesima, restringendo il dissenso a punti che assolutamente non definirei devastanti nella dialettica. Questo è un fatto importante, sul quale non speculo, e non sto a guardare la differenziazione preconcetta tra opposizione e maggioranza.

e cioè che l'avvocato non é un soggetto di impresa commerciale ed economica in senso proprio, né disciplinabile con le regole del mercato che vengono qui, quasi all'eccesso, sempre ricordate.

sbalorditive e rispettabili come tutte le posizioni. Ci mancherebbe altro che in un emiciclo non vi fossero estremismi contrapposti sul piano dialettico dei concetti, ma starei per dire, giocando banalmente sulle parole, che seguendo il andiamo su una pericolosa "ichina" di sregolatezza, di iperliberismo selvaggio: una disarticolazione auspicata e, direi quasi, un'anarco-demagogia. Non uso mezzi termini perché il suo estremismo, al di là della sua parola sempre ovattata e garbata, è in questi termini che deve essere qualificato. Ben diverso è l'atteggiamento del senatore Chiurazzi, il quale cerca di prendere le distanze da questo scempio dialettico a cui ho fatto riferimento e, pur criticando qualche punto, rivendica i fondamentali e, anzi, li fa propri.

di dire - non certo la capacità, ma la volontà di contrapporre delle linee ispiratrici alternative, che non ho sentito esporre. Una posizione più articolata e differenziata ci viene dal senatore Legnini, il quale tutto sommato contraddice la senatrice Della Monica su parecchi dei presupposti che la stessa ci ha illustrato, cercando di inserire alcune linee di possibile emendabilità,

Così come il senatore Galperti, pur dello stesso Gruppo del Partito Democratico, che tutto sommato ci ha dato assenso o consenso su quasi tutti i passaggi essenziali della riforma, restringendo alla questione del del sindacalismo giovanile quell'area di dissenso che il Partito Democratico evidentemente sta cercando di intestarsi nella sua libertà di manovra e di presa di posizione. di posizione. Dobbiamo affrontare il problema. Non, come oggi è di moda dire, in maniera non ideologica: a me non interessa se lo affrontiamo in modo ideologico o pragmatico, sono due estremismi di atteggiamento che mi carezzano poco. Andiamo all'essenziale, vediamo in cosa si traducono. Il Governo, invece, cui pure cui pure è stata mossa qualche critica questa mattina, si è contenuto bene e il ministro Alfano si sta confrontando con le categorie professionali, ha inaugurato una bella stagione di confronto, anche collegiale, sta rispettando il ruolo del Parlamento, e l'ha dimostrato anche oggi, in un corretto equilibrio che tutti, il Governo per parte sua e noi parlamentari, anche della maggioranza, dobbiamo rivendicare e garantire: un protagonismo del Parlamento nella dialettica, perché no, anche con l'Esecutivo, specialmente su argomenti come questo. Il Ministro ha mantenuto, però, l'impegno, che noi come maggioranza stiamo mantenendo, sull'urgenza di questo provvedimento, coerenti nel dimostrare che questo è un tassello essenziale di quella che, con parola troppo generica, viene chiamata riforma della giustizia, che significa tutto e non significa niente, se non si specifica in tasselli importanti e qualificanti, come questo indubbiamente è da noi considerato. Ecco perché vi ho detto, onorevoli colleghi, che il Popolo della Libertà, non in esclusiva, si intesta con forza e con convinzione questa riforma che, com'è stato detto, segue, dopo oltre settant'anni, la legge

ed è una legge che ha funzionato, eccome, per il semplice fatto che era fatta bene, era solida, mentre, nel tempo, non si è mai concretizzato un diffuso consenso delle categorie e dei ceti politici intorno ad un'ipotesi di riforma.

un ruolo, un posto e una voce, è favorevole all'impianto di questa riforma ed anche ai passaggi essenziali che attengono alla professione giovanile. Pertanto, fino a prova contraria, semmai le voci più consolidate vengono a corroborare l'impostazione di questo provvedimento.

consentitemi di dire, onorevoli colleghi di opposizione, che di certo noi non vogliamo quello che - ahimè! - nelle parole di molti di voi, voglio sperare non intenzionalmente, si vorrebbe.

dell'avvocatone con 30 avvocati e 125 praticanti nello studio? Questa è una visione propria anche di molti della sinistra: è impressionante, ma è così.

È dimostrato: non lo dicono solo gli avvocati. Ciò avviene in tutti i campi, ed anche nel settore della professione forense. Quindi, molti colleghi di opposizione finiscono per auspicare - voglio sperare inconsapevolmente - l'avvocatone - l'avvocatone o l'avvocatuccio. Abbiamo sentito - in qualche modo involontariamente - trapelare e trasudare dalle parole del senatore Legnini l'avvocatuccio, il giovane che cerca disperatamente di ritagliarsi un posticello nel ventaglio della professione, magari a tariffetta, con la causetta che si ripete con il ciclostile - egli dice - sotto il minimo: l'avvocatuccio proletario. Altro che visione di classe, collega Legnini! È lì la visione di classe: l'avvocatuccio proletario. Oppure l'avvocataccio, quello che si butta in pubblicità, che si organizza in un certo modo, che apre la bottega che affaccia sulla strada, quello che si mette a mezzi con il cliente, quello della quota lite, l'avvocataccio d'affari. Insomma, l'avvocatone, l'avvocatuccio o l'avvocataccio. E invece no. Tutto questo non è accettabile da parte nostra. Queste ipotetiche scelte - mi auguro involontarie - di taluni di voi si specificano poi in concreto.

settore. Qui no. Chiunque ha il pezzaccio di laurea in mano, prende ed entra in porta girevole, anzi, in porta a vento, come quella del *saloon* e poi, dopo, dentro il *saloon* avverrà la selezione del mercato.

persone, ma stiamo parlando di società di capitali, come se poi il capitale non condizionasse la libertà e le modalità di espletamento della professione.

anche perché, altrimenti, si dà luogo ai fenomeni del degrado e della prostituzione professionale. È esattamente questo quello cui mi riferivo prima. Chi non sa che oggi i grandi complessi economico-finanziari - in vari settori che non voglio star qui a dettagliare fanno i bandi? Chiamano il giovane alla disperata ricerca del guadagno di qualche carta da 100, dicendo: «Le vuoi le cause? Benissimo, allora sono 1.000 euro per ogni causa»: causona, causetta, causaccia, infondata o fondata. Mille euro! E quel poveretto che deve fare? L'avvocatuccio proletario, auspicato da alcuni di voi, accetta; e l'avvocato serio, allora? Le centinaia e le migliaia di avvocati seri e dignitosi che devono fare? Devono assistere a questo? È questo che chiedete? La quota lite? Non ci troviamo oltre Atlantico, è un'altra la tradizione istituzionale, culturale e professionale dell'Europa e, in particolare, italiana.

questo titolo così solenne. Apertura degli spazi professionali - altra linea coerente di molti oppositori - a coloro che non hanno titoli: si sta facendo strada questo discorso per cui tutti fanno tutto. tutti fanno tutto. Perché riservare spazi della professione all'avvocato, all'iscritto all'albo? Cos'è questo privilegio? No, tutti facciano tutto; si apra la bottega sulla strada del supermercato; si renda consulenza accessibile, immediata ed a buon mercato. Questo è nella linea della logica di alcuni di voi. Mi dispiace dirlo, colleghi; lo dico forse in maniera un po' colorita. Ciò vale anche per la libertà della pubblicità. Ma cosa è questo privilegio, paludamento? Ma chi credono di essere gli avvocati? Si fa la pubblicità ai dentifrici! La faccia anche l'avvocato! Come le massaggiatrici: si metta sui grandi quotidiani A.A.A massima riservatezza. L'avvocato si offre:

È nella vostra linea: siete coerenti, onorevoli colleghi, quando chiedete questo. Si vuole che i 12, i 15, i 22 praticanti dell'avvocatone rispunta il conflitto, senatore Legnini: non è classismo il nostro. Mi dispiace che proprio lei, che non credo sia un classista di cultura e di mentalità, si esprima in termini potenzialmente classisti. Voi volete 120 praticanti dello studione in conflitto sindacale con il barone dello studio o con i cinque baroni dello studio. Per un verso vi adeguate alla figura dei filmetti americani degli studi associati «Pinco & Pallino», «Johnson & Johnson» e per l'altro state parlando di una realtà che rischia di essere degradata se vi seguissimo su questa strada. Per questo vi dico che voi state andando, onorevoli oppositori, verso un avvocato che insistete quasi nel considerare non necessario. In questo, gentile rappresentante del Governo, qualche volta siamo un po' fiacchi concettualmente anche noi. Talvolta qualche breccia la apriamo indebitamente - e sbagliamo - nel considerare l'avvocato non necessario in certi passaggi. Per la conciliazione - altro fronte che «te lo raccomando» «te lo raccomando» - non è necessario l'avvocato. Quella è la fase più delicata dell'approccio al contraddittorio, al confronto tra gli interessi e le posizioni di diritti, eppure l'avvocato non è necessario. Veniamo prevedendo sempre più zone nelle quali l'avvocato non è necessario. Ciò mentre noi, avvocati più attenti, più evoluti, più avvertiti, cerchiamo di spiegare oggi modernamente - altro che causa più pende più rende! Qui parliamo allora dell'avvocato della coppia di capponi o della forma di formaggio dei primi del secolo, onorevoli colleghi

Quello che voglio precisare è che lei è stato informato che non c'era contingentamento dei tempi, ma questi sono i limiti posti dal Regolamento. *(PdL)*. Se lei non ritiene di ampliare la dotazione di tempo a mia disposizione, ancorché votazioni non vi siano e dagli uffici del mio Gruppo mi sia stata detta cosa inesatta, ne prendo atto, anche perché le mie parole non cambieranno la storia, non c'è dubbio: ragion per cui, penso che privarcene non sarà un fatto drammatico. Se però con la sua benevolenza mi concederà qualche secondo in più per tirare le mie conclusioni, vorrei dire che, di fronte a queste figure squallide e non condivisibili di avvocato che molti di voi descrivono, il Popolo della Libertà contrappone un avvocato degno di questo nome, soggetto costituzionalmente rilevante: avvocato capace, onesto, forte. Quando l'avvocato è forte e garantito in tale sua qualifica, la libertà è forte; quando l'avvocato è indebolito e proletarizzato, è la giustizia stessa che ne esce degradata. Ecco perché, concludendo - mi riservo eventualmente di depositare una nota scritta per l'illustrazione più diffusa degli argomenti che erano in serbo nel mio dire - siamo, come partito di maggioranza relativa, aperti ad un confronto su qualche singolo passaggio in cui il buonsenso e la funzionalità ci illuminino e ci consiglino al meglio, ma retromarce sono assolutamente escluse, perché la lunga attesa, il lungo confronto, la lunga maturazione e il lavorio di preparazione di una normativa di questo genere non giustificherebbero né rinvii né annacquamenti di identità.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia è una replica doverosa, perché nel corso del dibattito sono emersi più argomenti che meritano di essere presi in considerazione, che devono essere analizzati e che certamente non incidono sull'impianto generale del disegno di legge. Questo lo dico perché dico perché non ha subìto alcun *vulnus* il progetto che era stato preso in considerazione nel corso del lungo, puntuale e rigoroso impegno che il Comitato ristretto essere in Commissione giustizia, né sono emerse proposte che incidano radicalmente su quel testo, che poi la Commissione giustizia ha licenziato leggermente modificato rispetto a rispetto a quanto il Comitato ristretto non avesse fatto. Le proposte che sono venute dalla discussione sono tutte meritevoli di grande apprezzamento. Sono i temi su cui ci siamo confrontati e su cui continueremo a confrontarci nel corso del dibattito in Aula.

avvertiti intervenuti atteggiamenti di rottura, di categoricità rispetto all'impianto del disegno di legge. disegno di legge. È stato rimarcato egregiamente dal Ministro questa mattina che noi abbiamo cercato di uniformarci a quelle che erano le esigenze dell'avvocatura e della società.

Non basta essere avvocati, come molti di noi siamo, per conoscere a fondo i problemi complessi che si agitano all'interno della nostra categoria, nutrita da ben oltre 200.000 soggetti, in aree diverse del Paese. Quindi non basta la nostra esperienza; lo sapevamo, eravamo perfettamente consapevoli e ognuno di noi ha formulato delle proposte alla luce della propria esperienza, ma soprattutto abbiamo poi interloquito con le associazioni di categoria e con gli organismi istituzionali dell'avvocatura, qual è il Consiglio nazionale forense. Quindi, questo metodo lo rivendichiamo con orgoglio. Senatrice Poretti, non ci siamo fatti imporre dall'avvocatura le regole da riversare in questo documento legislativo, nel quadro di meccanismi, come dire, ideologici che vengono da lontano. No, noi abbiamo abbiamo adottato sistemi completamente diversi: è una legge che deve regolare la vita professionale degli avvocati; era inevitabile che discutessimo con gli avvocati. Spunti interessantissimi sono giunti dall'avvocatura, ma dall'avvocatura qualificata, da quella rappresentativa. Certamente non possiamo mettere insieme le esigenze sempre più complesse di 200.000 avvocati: ogni avvocato - soprattutto chi fa la professione lo sa - ha le proprie esigenze, le proprie pulsioni, è un soggetto che rivendica appieno la propria autonomia, questa è una peculiarità della libera professione. Mettere Mettere quindi insieme tutto sarebbe stato difficile; trovare soluzioni compatibili con tutte le plurime esigenze che l'avvocatura può rappresentare era un'operazione ardua: lo sapevamo bene, certamente non abbiamo coltivato nemmeno per un attimo l'illusione che tale obiettivo si potesse realizzare. Abbiamo però realizzato un documento legislativo che certamente le proposte e gli stimoli che vengono dall'Assemblea potranno migliorare; abbiamo realizzato un documento legislativo che scrive i momenti essenziali più utili e più moderni della vita professionale degli avvocati. Voglio replicare a qualche collega intervenuto che ha svolto pregevolmente argomenti a tutela delle proprie ragioni. Il senatore Carofiglio ha criticato tre momenti fondamentali di questo impianto legislativo: i criteri dell'accesso, la pubblicità e le tariffe.

altri l'hanno criticata *tout court* ed altri ancora hanno ritenuto che alcuni aggiustamenti potessero essere presi in considerazione. Condivido l'impianto emerso dalla discussione consentita l'espressione - più moderata e meno manichea, perché la materia oggi in esame esclude la possibilità di atteggiamenti di contrapposizione. non ci occupiamo di temi politici, ma discutiamo di come meglio regolamentare le funzioni e le attività di una categoria che ha un ruolo trainante nella vita del Paese

di rendere l'avvocatura assolutamente coerente con le esigenze ed i tempi che viviamo, non solo perché così viene reclamato dalla società, ma soprattutto perché

i suoi compiti, sta andando oltre, sta invadendo settori che certamente non possono essere attinti da quelle attività, a meno che non si realizzino momenti patologici. La verità è che registra un'imbarazzante invadenza di questo importantissimo organo, anche nella fase legislativa e soprattutto nella fase amministrativa. È importante, dunque, che vi sia un'avvocatura consapevole della propria funzione, determinata e documentata. cari colleghi, nasce l'esigenza dello studio costante, di un aggiornamento periodico, ma sistematico.

di documentarsi. La risposta è che se per venti anni si è retto alla concorrenza e alla competizione si è costituito un credito professionale e non vi è più bisogno di studiare per i venti anni successivi.

- quella dell'aggiornamento diventa solo una mia esigenza, perché non devo dimostrare niente a nessuno; non devo tutelare il consumatore, il quale, non avendo cognizione di chi sia il più bravo o il meno bravo

hanno sollevato il problema della criticità con cui l'*Antitrust* sta considerando il nostro impegno e la nostra fatica. i meccanismi del mercato impongono regole particolari per cui l'offerta può essere anche al ribasso, perché è così che la concorrenza si alimenta.

non si possano soltanto proporre soluzioni in termini economicamente più contenuti rispetto all'antagonista o al rivale professionale: i professionisti debbono proporre qualità. Quindi, una legge deve porre tutti in condizione di attingere alle fonti della qualità, anche se poi naturalmente le dinamiche interne della vita professionale, i rapporti, i successi e le contrapposizioni utili creeranno il soggetto particolare al quale si rivolgerà il cliente, l'assistito. A questo proposito, onorevoli colleghi, voglio ricordare quanto è stato scritto da un illustre giurista, un grande civilista, Antonino Cataudella, titolare della cattedra di diritto civile all'Università di Roma, in una monografia contenuta nella «Rassegna di diritto civile». civile». Il tema trattato è più vasto, ma egli scrive qualcosa a proposito di quelle che, in maniera gergale, furono chiamate le lenzuolate di Bersani: «Avere esclusivo riguardo all'incentivazione della concorrenza in questi settori significa, se la finalità della concorrenza resta esclusivamente mirata all'abbassamento dei corrispettivi, disattendere l'esigenza primaria del consumatore, che è quella di poter scegliere un professionista qualitativamente adatto al compito che intende affidargli». Egli dice in mirabile sintesi, con l'essenzialità del grande giurista, le cose che io in maniera un po' più enfatica ho detto poc'anzi. Aggiungo anche

come riferimento normativo cui uniformarci ogni qualvolta ci avviamo a modifiche che incidono su settori sensibili della vita del nostro Paese - e l'avvocatura certamente lo è

attenta e priva di preconcetti, hanno escluso che un sistema tariffario quale quello esistente in Italia prima della legge Bersani fosse contrario alle regole di concorrenza. Ecco allora che gli argomenti pregevolmente introdotti dal senatore Carofiglio e da altri colleghi

sopravviene però la meditazione successiva, *melius re perpensa*, la lettura dei testi dattiloscritti ed emerge il dato sul quale si deve appuntare la critica, se si deve appuntare. Su un passaggio fondamentale

In tema di incompatibilità abbiamo realizzato una compiuta osservazione, ci siamo interrogati con con autorevoli colleghi dell'opposizione e abbiamo individuato quali debbano essere le incompatibilità, cioè quelle attività che si pongono su un piano assolutamente divaricato rispetto all'attività dell'avvocato, quando sussiste una difficoltà oggettiva

certo clima di demagogia abbia permeato le parole del collega Maritati, che si dica che l'attività di parlamentare

la disponibilità ad una discussione ulteriore che certamente in quest'Aula ci sarà. Lei ha detto che nel momento in cui

di un sistema paritario organizzato all'interno di strutture societarie e associative, sussistono tutte le condizioni perché l'impianto normativo, di cui oggi stiamo discutendo, possa considerarsi aderente alle esigenze dell'avvocatura.

un fondo spese al giovane collaboratore la discutemmo ampiamente, giungendo ad una conclusione. Molti avvocati

se non vi è quest'obbligo - praticare uno studio, conoscere gli ambienti dell'avvocatura e lì costituire magari rapporti forieri di un trattamento economico diverso, soddisfacente. Abbiamo pensato che, se imponiamo l'obbligo del conferimento del pagamento di un fondo spese, del riconoscimento di una piccola somma, potremmo creare delle difficoltà all'accesso; però non abbiamo inibito la possibilità non abbiamo inibito la possibilità che i giovani, nel momento, difficile ed impegnativo, del tirocinio, svolgano altre attività private. private. Noi abbiamo escluso il concorso pubblico, perché se si fa l'impiegato al Ministero non si può fare il praticante avvocato. Ho sentito dire da qualche collega che vi era una sorta di iato insuperabile fra qualsivoglia tipo di attività ed il tirocinio. Non è così:

ad individuare soluzioni che risolvano questo problema. Resta ferma, naturalmente, l'inibizione rispetto allo svolgimento di compiti presso le pubbliche amministrazioni.

la professione rispetto a quei consessi, a volte prestigiosissimi, a volte ineffabili, che propongono tutela giudiziaria, che propongono pareri legali, ma che non hanno i titoli.

vuole, non è compatibile con le esigenze più avvertite di coloro che debbono fruire dell'attività di patrocinio di un avvocato.

lui avanzate sono tutte meritevoli di attenzione. Io, però, ho un atteggiamento di assoluta fermezza in ordine ai minimi tariffari; le determinazioni cui giungerà l'Assemblea sono come sempre sovrane. Non si tutelano i giovani, senatore Legnini, nel momento in cui si consente un'eccessiva dinamica nel mercato per cui si possa proporre qualunque soluzione economica e si costituisca una sorta di offerta al ribasso. Abbiamo assistito - e mirabilmente ne ha parlato Antonino Caruso - all'atteggiamento adottato dalle grandi strutture che si avvalgono della consulenza professionale e dell'opera di professionisti. Nella piena consapevolezza che esse sono un interlocutore privilegiato per qualunque avvocato, salvo coloro che non rinunciano alla dignità e quindi ai mandati (perché questo accade ed è accaduto) si manda un tariffario modestissimo in cui si prevede - e la più parte di questi clienti così fanno - che, qualunque sia l'entità della causa e la sua difficoltà, se si vuole avere un rapporto continuativo, gli onorari non possono superare quelli relativi ad una causa che abbia un valore inferiore a 500.000 euro.

che l'impegno professionale di un avvocato deve essere valutato per quello che è; poi, le regole antiche

a conclusione del suo intervento, che il disegno di legge in esame, con i temperamenti, le modifiche e i cambiamenti che il Senato riterrà necessari, ma nella solidità del suo impianto di base, possa essere approvato entro i tempi più brevi possibili. *(Applausi

Signor Presidente, svolgerò alcune brevi considerazioni, essendo già intervenuto autorevolmente il Ministro. La relazione, la discussione e la replica del relatore hanno già illustrato i contenuti e gli aspetti di questa importante riforma, che giunge all'esame dell'Assemblea di Palazzo Madama. Non c'è bisogno che aggiunga altro sul merito, perché ciò che è stato evidenziato con passione e competenza è il risultato di un lavoro attento, paziente e partecipato che ha definito scelte di equilibrio difficili, adottate tra esigenze talvolta anche contrapposte, ma sempre nella consapevolezza dell'impossibilità di lasciare una professione come l'avvocatura in un sistema come quello della giustizia italiana senza un convinto intervento di ammodernamento. Come rappresentante del Governo, tuttavia, vorrei considerare brevemente tre aspetti di questa riforma, particolarmente degni di attenzione: il metodo, l'ispirazione e le finalità. Quanto al metodo, e su questo aspetto si è anche soffermato il senatore Valentino, è importante ribadire come tra i molti meriti di questa riforma c'è proprio quello di un *modus procedendi* continuativamente improntato al più ampio coinvolgimento. Fin dall'inizio, infatti, il testo si è giovato di un concorso determinante proveniente dall'interno delle articolazioni rappresentative del mondo forense, che erano state espressamente invitate dal Ministro all'apertura della legislatura ad elaborare una proposta unitaria. Successivamente, l'esame parlamentare è stata svolto in un clima costruttivo e competente che ha visto un fondamentale apporto di tutte le componenti politiche, oltre che della dedizione del relatore, che ha significativamente ricordato il ruolo del senatore Calvi nel corso delle passate legislature. Questa riforma è attesa da un numero di anni che, come tutti bene sapete, sorpassa di alcune decadi le responsabilità di questo Governo. Il confronto tra parlamentari, Esecutivo ed avvocatura in compenso è stato negli anni della legislatura in corso continuo, come continua è stata la presenza e l'adesione del Governo che non ha fatto mancare la massima attenzione nel dibattito, valorizzando i numerosi e preziosi spunti emersi, non sempre con identità di vedute. Il Governo è, tuttavia, ben consapevole dei meriti collettivi che si sono trasfusi nel testo al nostro esame, e ringrazia sinceramente tutti coloro che hanno così validamente presieduto, guidato ed arricchito il dibattito. Vorrei poi sottolineare il tratto di questo testo, perché ha, ad avviso del Governo, quella ispirazione che caratterizza le riforme che veramente servono al Paese. Il Governo non considera dignità e prestigio delle professioni come valori incompatibili con gli interessi del singolo cittadino, come se un intervento regolatore non possa che considerarli in relazione inversa ed aggiungere all'uno necessariamente sottraendo all'altro. Non c'è nulla di più infondato. Si tratta di valori che si rafforzano insieme e che la riforma coerentemente e giustamente persegue entrambi. Non è inelegante - concordo con il collega relatore, senatore Valentino - ricordare invece quello che la filosofia della riforma espelle, vale a dire quel tratto punitivo che improvvidamente è stato talvolta il marchio della legislazione passata nei confronti delle professioni, sull'errato presupposto che l'interesse del cittadino si rafforzi solo di fronte all'arretramento del ruolo del professionista. Non è questa il metodo e non è questo il fine. Quanto alla finalità, invece, si tratta pur sempre di dare compiuta ed aggiornata attuazione a precetti di rango costituzionale.

davanti a un giudice terzo entro una ragionevole durata. La riforma forense è un architrave per costruire un sistema di giustizia capace di assicurare concretamente e durevolmente questi valori. L'avvocatura - questo è il nostro convincimento - deve essere messa in condizioni di operare al meglio, con un rango ed un'attenzione pari a quello della magistratura. L'Esecutivo ha sempre avuto piena consapevolezza del ruolo cruciale che le professioni forensi svolgono all'interno dei delicati e complessi meccanismi di funzionamento della macchina processuale ed è stato sempre assolutamente convinto che nessuna riforma, né del rito civile né di quello penale, potrà raggiungere gli obiettivi che si propone non solo contro, ma neppure senza o anche solo sopra le categorie professionali che della giurisdizione sono elemento primario di evidentissimo rilievo. Questi concetti sono stati autorevolmente confortati dai recenti interventi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Senato in occasione delle iniziative per l'inaugurazione dell'anno forense lo scorso 10 marzo. Quella che oggi il Governo invita ad approvare in modo convinto non è una riforma di settore, ma un contributo all'ammodernamento di una professione che opera in una società complessa e in un mercato globale, chiamata a dare un apporto fondamentale alla riuscita di un'operazione tanto complessa e delicata quanto indilazionabile e doverosa: l'uscita della funzione giurisdizionale dalle attuali condizioni di emergenza per dare al Paese quel sistema giudiziario equilibrato ed efficiente che merita.

Signor Presidente, colleghi, prendo la parola per ricordare nell'Aula del Senato che sabato prossimo, il 24 aprile, ricorre il 95o anniversario di ciò che il popolo armeno considera l'inizio del grande male, «Medz Yeghern», dello sterminio razziale, come lo definì allora l'ambasciatore americano presso in definitiva del genocidio degli armeni quando, nel 1915, nell'Impero ottomano fu consumata l'azione mirata all'eliminazione degli armeni presenti su quel territorio.

nella convinzione che il suo comune riconoscimento possa costituire la base per nuovi e duraturi rapporti di collaborazione tra la Turchia e l'Armenia, previsti del resto dal recente storico accordo, firmato a Zurigo il 10 ottobre 2009, di normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi, tra due Repubbliche decisive nell'area tra l'Unione europea e il Medio Oriente, culla di antiche civiltà chiamate oggi a costruire progresso e pace per tutti, nel riconoscimento dei diritti umani universali e dei crimini contro l'umanità. La memoria del massacro degli armeni, che aprì nella vergogna il XX secolo, che fu chiamato il secolo dei genocidi, ci sollecita oggi a lavorare sia perché il Senato della Repubblica italiana si pronunci presto sul riconoscimento del genocidio, sia perché si realizzi, un secolo dopo, la grande riconciliazione, che non è soltanto tra Turchia e Armenia, ma è parte della stessa vita dell'Europa, sulla base della verità storica, verità che noi oggi consideriamo come parte della nostra comune memoria europea.

Uno dei capitoli di questo accordo affronta la questione testé citata, e che verrà ricordata sabato prossimo. Si è deciso, tra l'altro, di adottare un approccio simile a quello che l'Italia, in passato, ha adottato con la Slovenia, relativamente ad altri eccidi avvenuti in passato.

in virtù di questa ispirazione che è alla base dell'Unione europea - che magari negli ultimi anni si è distratta dai propri principi fondativi - credo che si debba fare quanto più possibile perché tra le parti si riesca a trovare

affrontare la questione e perseguire un risultato che possa avere, alla fine del percorso intrapreso, l'obiettivo di consegnare alla storia ciò che è avvenuto, e guardare avanti. Credo che, come è avvenuto in alcune Assemblee legislative, da ultimo nel Congresso degli Stati Uniti, imporre la la pronuncia da parte di una delle due Camere, o di tutte e due, relativamente alla richiesta di dover riconoscere quel che è avvenuto in passato, che appartiene non soltanto al passato ma anche a regimi passati, non vada necessariamente nella direzione del guardare avanti per trovare soluzioni. Sono ormai più di due anni che l'Europa e gli Stati membri dell'Unione europea non fanno niente per aiutare l'ingresso della Turchia, e magari, perché no, anche dell'Armenia nell'Unione. Credo che l'iniziativa che si cerca di portare avanti con una mozione che chiederebbe al nostro Senato di esigere il riconoscimento dei fatti del secolo scorso non vada nella direzione auspicata dell'aiuto a chi ha dimostrato - quello sì - negli ultimi cinque o sei anni

luglio 2008. Faccio riferimento alla legge n. 157 del 1992, che prevede la possibilità per le Regioni di autorizzare la cattura di uccelli ai fini di richiamo tramite l'attivazione di impianti speciali.

qualificato, con licenza particolare, ritenuto idoneo da quello che è stato l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Molti tra i gestori dei roccoli sono anche i proprietari di detti impianti e li tengono come veri e propri giardini nelle nostre Prealpi e Alpi italiane. In Lombardia, in particolare, l'età anagrafica avanzata di detti gestori pone un problema di ricambio generazionale. Sia la Provincia di Bergamo, sia la Regione Lombardia hanno fatto specifica richiesta all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, oggi ISPRA, per indire concorsi specifici a rilasciare le autorizzazioni al prelievo di questi uccelli in deroga. Sia alla Provincia bergamasca, sia alla Regione Lombardia è stato risposto picche, cioè che non sono in grado di autorizzare o di fare questi nuovi esami. Considerato che proprio in questi giorni alla Camera si sta discutendo sul mantenimento vediamo innanzitutto di far funzionare questi enti. Diversamente è inutile che in Parlamento stiamo a discutere di enti che non funzionano, discussioni che si riducono a scaramucce parlamentari, mentre non riusciamo a far progredire ed avanzare determinate leggi.

È difficile, per la verità, avere dal Governo delle risposte agli atti di sindacato ispettivo, ma io, come rappresentante unica del movimento Io Sud nell'ambito del Gruppo al quale appartengo, ritengo che d'ora in poi questa assise debba interessarsi realmente dei problemi del Mezzogiorno, che non devono rimanere affidati soltanto soltanto ad uno sterile dibattito giornalistico. Tutti vogliono interessarsi del Mezzogiorno, ma nel momento in cui si cerca di individuare alcune soluzioni nessuno intende affrontarle nella sede opportuna, che è appunto quella parlamentare. Di fatto si sta attuando un federalismo, che è quello fiscale, indubbiamente, ma che è la forma peggiore di federalismo, che ci porterà ad una secessione, che qualcuno definiva dolce qualche tempo addietro e che io ritengo ormai una secessione di fatto, tra una macroregione del Nord, che diventerà sempre più ricca, e le Regioni del Sud, che diventeranno sempre più povere. Il mio atto di sindacato ispettivo riguarda la graduatoria delle università italiane, che ha visto una forte penalizzazione di tutte le università del Mezzogiorno d'Italia. Si chiede al Ministro di partecipare attivamente all'attuazione del federalismo, consentendo a

dalla stessa linea di partenza; altrimenti il federalismo diventa penalizzante piuttosto che propositivo, attivo e di sana competitività fra i territori. Le chiedo perciò, Presidente, di intervenire presso il ministro Gelmini perché ci dica se ha intenzione o meno di rivedere i parametri, che attualmente sono fortemente penalizzanti per tutte le università del Mezzogiorno.

ad unanimi decisioni rispetto a linee d'indirizzo meno penalizzanti per le università del Sud. Presidente, vorrei intervenire su quanto detto dalla senatrice Soliani, e anch'io - come il collega Perduca - lo faccio da amico della Turchia. Presidente, ci sono fatti su cui la politica ha diritto di intervenire, ma ci sono anche vicende su cui la politica ha il dovere di lasciar fare agli storici. Mi riferisco a vicende controverse come, ad esempio, quella dell'eccidio degli armeni, che gli armeni definiscono genocidio, collega Soliani, ma che i turchi rifiutano di definire in tal modo. Essi sostengono infatti che se eccidio ci fu - molti storici turchi lo riconoscono, e c'è un dibattito acceso e forte nella comunità degli storici e degli e degli intellettuali turchi in questo senso - non si può assolutamente parlare di genocidio, perché non c'era l'intento di sterminare un'etnia, e non ci fu programmazione del massacro. massacro. Nella società turca, nelle università turche, tra gli intellettuali turchi è in atto un dibattito interessantissimo, che dobbiamo seguire con grande rispetto,

e non c'è peggior danno che si possa fare al processo di riavvicinamento e di riappacificazione tra la Turchia e l'Armenia che insistere su questo argomento e pretendere dall'esterno che i turchi operino un riconoscimento di un fatto contestato anche dal punto di vista storiografico. Vi è una città turca, vicino ai confini dell'Armenia e molto vicino al monte Ararat, dove c'è una stele che ricorda il massacro che gli armeni hanno fatto di centinaia di migliaia di turchi. La storia di quella regione è perciò contrastata,

verrebbe percepito come una forzatura ed un'intromissione nella sua

come è accaduto, l'Unione europea ha anche accantonato la priorità del riconoscimento del genocidio come *conditio sine qua non* per l'ammissione della Turchia.

il rapporto annuale, in questo caso relativo al 2009, sui lineamenti di politica del Governo in materia di controllo delle esportazioni e delle importazioni e del transito dei materiali di armamento. Non si parla di armi di piccolo calibro, ancorché usate sicuramente molto nei tanti conflitti a bassa intensità che ci sono nel mondo, ma si parla proprio di armamenti. La legge n. 185, che viene reputata una buona legge anche a livello internazionale, è buona anche proprio per questa trasparenza e per questo rapporto che annualmente il Governo ogni anno deve fare sul transito dei materiali di armamento. Peccato che quest'anno il rapporto fatto dal Presidente del Consiglio dei ministri il 29 marzo 2010 manchi di un allegato importante, quello che riporta l'indicazione delle singole operazioni autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze agli istituti di credito, relative proprio all'esportazione delle armi italiane,

si vedono quindi quali banche hanno autorizzato, quali banche sono intervenute e quali no. È previsto dalla legge ed è un elenco importantissimo, perché permette alla società civile, ai singoli correntisti interessati ai temi della responsabilità sociale di impresa e delle dichiarazioni etiche, di verificare se effettivamente effettivamente le direttive e le intenzioni emanate negli ultimi anni da diversi ed importanti istituti di credito italiani in relazione ai servizi d'appoggio e al commercio di armi sono effettivamente attuate; credo quindi sia importante conoscere anche questo allegato. Pertanto, nell'interpellanza chiedevamo perché mancasse questo allegato

che noi addirittura abbiamo giudicato estorsivo da parte di Equitalia, della Gerit, degli altri concessionari che

di Commissione finanze abbiamo chiesto l'audizione dei vertici della società, perché, lo ripeto, la Corte di cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 407 del 2010, ha sancito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per un importo inferiore a 8000 euro. Richiedere tributi prescritti e inviare cartelle esattoriali non dovute, oltre a mettere in moto un meccanismo perverso, in aperta violazione dello Statuto dei diritti dei contribuenti, impone al cittadino l'inizio di una vera e propria *via crucis,* con perdite di intere giornate lavorative ripeto - configurando addirittura il reato di estorsione quando per piccoli importi di qualche centinaio di euro il contribuente si vede costretto a pagare due volte, piuttosto che avviare l'onerosa pratica fatta di code interminabili presso gli uffici di Equitalia dove poter effettuare la contestazione. Se non si rispettano i diritti, soprattutto dei cittadini, dei pensionati, di coloro che magari sono stati multati anche con la tecnica degli agguati, significa che